L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 29 maggio 2018 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze* «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, la discussione in Aula e i diversi interventi delle forze politiche hanno espresso apprezzamento per il valido lavoro svolto dalla Commissione speciale, a dimostrazione del fatto che il Parlamento ha mostrato interesse ad affrontare la questione Alitalia. La necessità di colmare il vuoto informativo ha indotto, in sede di Commissione speciale, a richiedere e ad avviare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, grazie anche al sostegno di tutti i Gruppi parlamentari, un'indagine conoscitiva

oltre alle criticità gestionali delle precedenti amministrazioni che si sono succedute, le tante difficoltà ancora da superare. Nonostante i primi risultati ottenuti, peraltro dai valori contrastanti, il risultato economico finale del periodo commissariale da maggio a dicembre 2017 si chiude infatti con una perdita di 160 milioni di euro, senza considerare gli alti oneri finanziari, le partite non ricorrenti e le imposte. Con riferimento ai finanziamenti concessi oggetto del presente procedimento in esame, l'indagine conoscitiva ha anche permesso di appurare che, alla data del 30 aprile 2018, il saldo di cassa è pari a soli 769 milioni di euro, insufficiente a garantire non solo il rimborso del prestito e degli interessi maturati, ma anche la stessa sopravvivenza prossima di Alitalia. Il tempo, pertanto, per scongiurare l'ennesimo fallimento è molto ridotto. Il conciso e proficuo dibattito, prima in Commissione speciale e dopo in Assemblea, ha rilevato la pressante, avvertita e urgente necessità di risolvere questa importante vertenza nazionale che risulta legata a quattro aspetti fondamentali. Innanzitutto, vi è l'eventuale processo di vendita di cui già si parla da tempo e per cui fondamentale sarà la scelta di soggetti acquirenti per non disperdere un importante *asset* strategico del Paese. In secondo luogo, c'è la ricerca di nuovi investitori capaci di garantire quelle risorse fondamentali per consentire ad Alitalia di possedere una solidità patrimoniale in grado di riacquistare il mercato di lungo raggio maggiormente redditizio. la redazione di un piano industriale che sappia garantire razionalità nei costi e una gestione profittevole. un *management* altamente professionale e privo di conflitto di interessi che sappia garantire economicità, solidità a tutta l'organizzazione aziendale e condivisione con gli obiettivi di puro benessere collettivo. Sarà, pertanto, compito del nuovo Governo, legittimato nei suoi poteri, a porre tra i temi centrali del dibattito politico il tema in discussione e a programmare il rilancio - si spera definitivo - dell'ancora amata e sentita compagnia di bandiera. Il tempo a disposizione non è tanto e, in caso di mancate soluzioni tempestive, sarà inevitabile assistere all'ennesimo fallimento, da cui conseguirebbero gravi e incontrollabili problemi occupazionali, sociali ed economici. Prima di concludere sento la necessità di ringraziare il funzionario della Commissione speciale sugli atti urgenti del Governo, nella persona del dottor Alessandro Goracci, e tutti i suoi collaboratori per il supporto e l'eccellente lavoro svolto nel corso dell'esame di questo decreto-legge, così come di tutti gli altri provvedimenti assegnati alla medesima Commissione. Un ringraziamento particolare, infine, è doveroso rivolgere al Presidente della Commissione speciale, senatore Vito Crimi, e a tutto l'Ufficio di Presidenza per il lavoro profuso, nonché ai colleghi senatori che hanno esaminato e migliorato il provvedimento in esame.*(Applausi dal Gruppo M5S)*.

agli articoli del decreto-legge da convertire. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, come modificato dalla recente riforma, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno presentati ad un articolo si svolge un'unica discussione. In sede di illustrazione potrà intervenire un solo rappresentante per Gruppo, per cinque minuti. Per ciascun Gruppo è ammesso inoltre l'intervento di un ulteriore senatore, per non più di cinque minuti. Vorrei ricordare a tutti che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, è da oggi operativo il sistema di voto da postazione fissa. Invito pertanto ciascun collega a votare dalla propria postazione. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del

L'emendamento che abbiamo presentato e che vorrei illustrare era stato già presentato in Commissione speciale per gli atti urgenti del Governo, ma purtroppo in quella sede non era stato approvato, motivo per il quale Fratelli d'Italia ha deciso di ripresentarlo in Aula. In sostanza, occorre considerare che non è possibile parlare del vettore nazionale Alitalia senza parlare anche della rete aeroportuale. Come in tutto ciò che riguarda il sistema Paese, in teoria, prima si fa la strategia sulle reti - vale come esempio per quel che riguarda il trasporto ferroviario - e poi si parla dell'eventuale servizio fatto su quella rete: il sistema ferroviario italiano prevede RFI, a proprietà pubblica, e poi una concorrenza fatta dai vettori su quella rete pubblica.

*(FdI)*. L'ordine del giorno che abbiamo presentato, in sostanza, pone l'accento sulla necessità di parlare anche del sistema aeroportuale: parlare di Alitalia senza farlo del sistema aeroportuale è - a nostro avviso - un errore. In particolare, già lo studio One Works

il cambiamento non è da poco anche per Alitalia. Il Piano del 2012 prevedeva, infatti, che l'aeroporto di Fiumicino fosse destinato prevalentemente al trasporto di lungo raggio, diventando di fatto «casa Alitalia», e che le compagnie *low cost* dislocate in un terzo aeroporto del Lazio. Questo terzo aeroporto del Lazio nel piano aeroporti del 2014 è stato eliminato, senza spiegare come sarebbe riorganizzato il trasporto aereo a livello nazionale su Fiumicino né cosa sarebbe stato di Alitalia. Questo è il motivo per il quale oggi, nell'ordine del giorno che presentiamo, chiediamo al Governo ridiscutere del Piano nazionale aeroporti; in particolare per quanto riguarda Fiumicino, tornare a ragionare sull'ipotesi iniziale del 2010 - confermata da ENAC nel 2012 e riconfermata dal Governo addirittura nel luglio del 2013 - che prevedeva un piano aeroporti che includesse il terzo aeroporto del Lazio; conseguentemente, bloccare l'inutile speculazione sull'aeroporto di Fiumicino, con un raddoppio del sedime aeroportuale che non ha alcun senso. L'ordine del giorno impegna, quindi, il Governo a rivedere il piano nazionale aeroporti e prevedere un potenziamento dell'aeroporto di Fiumicino all'interno dell'attuale sedime aeroportuale. Si chiese tutto questo perché, in una grande fase di confusione della strategia sul trasporto aereo, ci ritroviamo - senza che nessuno abbia ben capito né come né chi lo abbia deciso - con un piano completamente diverso che penalizza l'Italia, la quale si trova ad avere sul proprio aeroporto di riferimento anche le compagnie *low cost*, e con un raddoppio del sedime aeroportuale di Fiumicino che penalizza la stessa città di Fiumicino e non ha alcun senso di logica aeroportuale.

anche se non appare proprio condivisibile la premessa, nella parte in cui si afferma testualmente che «l'incertezza politica venutasi a creare dopo le elezioni del 4 marzo 2018 ha frenato i possibili investitori a definire offerte adeguate, causando un rallentamento della procedura ed impedendo

Senatore Ferrari, da un punto di vista tecnico è prevista la possibilità per il relatore di presentare emendamenti e ordini del giorno in Assemblea, anche nel corso dei lavori, nonché di procedere a riformulazioni,

con l'auspicio che per la compagnia di bandiera possa aprirsi una fase nuova, con l'ingresso di soggetti che sappiano valorizzarne le potenzialità e chiudere finalmente la fase della gestione commissariale e dei finanziamenti ponte da parte dello Stato. L'importanza di Alitalia rispetto agli interessi del Paese non si può mettere in discussione. Inoltre, l'aumento dei passeggeri e dei ricavi nel primo semestre di quest'anno son la riprova delle potenzialità della compagnia, purché purché alla base vi siano una gestione oculata e la costruzione di un'offerta qualificata per i passeggeri nazionali e internazionali. L'auspicio è che i potenziali acquirenti sappiano farsene carico attraverso la salvaguardia dei posti di lavoro. Per quel che riguarda le modifiche apportate in Commissione speciale, il nostro Gruppo, rappresentato dal senatore Laniece, si è astenuto. Riteniamo infatti che, se - da un lato - vi è la necessità di acquisire con maggiore frequenza elementi informativi sulla situazione di Alitalia, dall'altro si rischia di lanciare un messaggio negativo sulla gestione commissariale, che invece - come i dati di questo semestre dimostrano - sta interpretando interpretando il proprio ruolo in maniera positiva. Si tratta di un aspetto delicato, anche in virtù delle indagini della procura di Civitavecchia, che ha acceso una luce sinistra sui 400 milioni di buco risalenti al primo anno di gestione Ethiad e sulla cessione a quest'ultima di *slot* particolarmente pregiati. Toccherà al nuovo Governo seguire con particolare attenzione l'evolversi delle trattative, nella speranza che si possa finalmente chiudere una situazione di travaglio che dura ormai da troppi anni. Ed è con questo auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in

è assolutamente importante, anche se riguarda semplicemente il differimento al 31 ottobre 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di gara. di gara. Vorrei ricordare che con questo decreto-legge si procede a una proroga fino al 15 dicembre 2018 della durata del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, che era stato già

industriale ed in questo caso anche sulla nostra compagnia di bandiera. La vicenda dell'Alitalia, con un aggravamento delle condizioni complessive di crisi nell'ultimo biennio, rappresenta esattamente e plasticamente - oserei dire - proprio il

dopo l'istanza depositata il 2 maggio dalla società stessa, nella quale si evidenziava una situazione patrimoniale assolutamente drammatica dal punto di vista dell'esposizione debitoria.

il quale i dipendenti di Alitalia bocciarono sonoramente il verbale di accordo stipulato il 13 aprile 2017 tra il Governo,

focalizzato solo ed unicamente sul taglio del costo del lavoro, che oggi è molto più basso - vorrei ricordarlo ai principali concorrenti nel settore. Tra l'altro, quel piano era centrato principalmente sul risparmio di breve periodo, prima degli investimenti necessari per il rilancio della compagnia. Ancora una volta sacrifici da una parte sola: mentre in meno di dieci anni i lavoratori di sacrifici ne hanno fatti molti, manca ancora una volta un vero e proprio piano industriale di rilancio e di investimenti che sia minimamente credibile. Noi non possiamo assolutamente considerare, quindi, il fallimento dell'azienda dell'azienda Alitalia come un destino ineluttabile: si può agire, si può rilanciarla, si possono fare scelte strategiche diverse, si possono ridare una storia e un decoro ad

che escluda qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o, ancora una volta, di spezzatino della compagnia e che possa invece rilanciare con forza la prospettiva. Noi pensiamo - e lo abbiamo espresso con un ordine del giorno che è stato tra l'altro approvato, anche se con la formula

molto serio. Riteniamo che questa iniziativa sia indispensabile per promuovere il rilancio di Alitalia e garantire l'integrità dell'insieme delle attività svolte. Quindi bisogna tenere insieme Alitalia e non accettare lo spezzatino. Il secondo elemento riguarda il fatto che la situazione la situazione di Alitalia, che ha condotto il Governo alla scelta dell'amministrazione straordinaria, è da molti anni così critica a causa di gravi errori di amministratori e dirigenti. Sono stati solo errori?

che il *management* non ha intaccato, salvo - ancora una volta - scaricare sui lavoratori (poi andiamo a vedere i loro *bonus* e le liquidazioni). Infine, penso anche all'attuazione inspiegabile di una strategia di ridimensionamento aziendale senza alcun intervento efficace

Inoltre, era prevista l'accessibilità da parte degli interessati alle informazioni sulle cause dell'insolvenza attraverso la pubblicazione di una relazione, che però non fornisce affatto

e poc'anzi in Assemblea, per richiedere ai commissari una relazione esaustiva sulle azioni degli amministratori che consenta, appunto, di accertare le ragioni e, quindi, promuovere le conseguenti ed eventuali azioni di responsabilità. Si tratta di una questione di serietà e trasparenza

non sfugge a nessuno che questo sia il primo provvedimento della nuova legislatura che giunge in Aula. Non vorremmo che che il provvedimento riguardante l'Alitalia

il simbolo e l'emblema di un Paese in stato di necessità. Che l'Alitalia sia in stato di necessità è dimostrato anche dall'imbarazzo del Governo in carica, in carica, ancorché solo per l'ordinaria amministrazione, di fronte al provvedimento in esame. Un Governo che si fa fregio di rispettare le regole europee,

un'ulteriore proroga che, di fatto, porterebbe la gestione commissariale e il prestito a ben valicare i termini europei

Parlo di un Governo che si faceva fregio di rispettare le regole europee e che ci consegna ora un provvedimento e un'Alitalia con un prezzo di 900 milioni, non più già allo stato dei fatti restituibile con gli interessi del 10 per cento che maturano ogni giorno, non indifferenti,

sia per la durata del prestito, che non avrebbe dovuto superare i sei mesi (mentre qui siamo a oltre dodici e alla richiesta di altri sei), sia per quanto riguarda la consistenza dell'aiuto, che la Commissione ritiene superare il limite minimo necessario. Questa indagine della Commissione è stata annunciata il 23 aprile. Dopo che la Commissione annuncia un'indagine per aver già valicato, a parere della Commissione, il tempo massimo necessario e concedibile e anche l'importo massimo necessario e concedibile, il Governo in carica, che si fregia di essere europeo, proroga di altri sei mesi. Come a dire: vi firmiamo per l'accertamento, ci fate vedere i documenti e, nel frattempo, noi continuiamo a operare. Io credo che questa sia una bomba ad orologeria, che può esplodere nei prossimi mesi (ancorché ci auguriamo che non accada), lasciata al prossimo Governo incaricato e legittimato dal nostro Parlamento. La seconda questione su cui vorrei far riflettere i parlamentari è che la gestione commissariale è iniziata oltre un anno fa. una cosa, al di là del giudizio che ciascuno di noi può dare, alla luce anche dell'indagine conoscitiva giustamente avviata dalla Commissione (perché quello che sta emergendo va portato alla luce in Parlamento e anche nel Paese). Benissimo, i commissari hanno iniziato l'attività oltre un anno fa: siamo alla seconda proroga, quindi al terzo mandato semestrale. Cosa è stato fatto in questo periodo per raggiungere l'obiettivo di vendere l'Alitalia a qualcheduno che magari ci conceda di avere ancora un vettore nazionale?

europeista, in questo caso viola in maniera conclamata e ripetuta le regole europee, con il rischio che poi pagheremo ovviamente i costi di questa violazione? Cosa ha fatto un Governo che appare decisionista nella politica industriale, per raggiungere l'obiettivo che si era posto con il primo provvedimento di oltre un anno fa e con il commissariamento, cioè la vendita di Alitalia? E perché la vendita di Alitalia non è stata fatta in questo periodo, in una condizione ottimale sul piano internazionale? Tutti noi sappiamo che una delle condizioni fondamentali perché un vettore possa stare in campo è rappresentata dal prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio, fino a qualche settimana fa, era ai suoi minimi.

non si sono create le condizioni per vendere l'Alitalia in questo anno, quando le condizioni erano migliori sul mercato del petrolio, come si farà a venderla nei prossimi mesi, entro la fine di ottobre? Basterà la terza proroga o ci vorrà la quarta?

un anno e mezzo in più li rende ancora più vecchi: quindi essi hanno ancora minor valore rispetto ad un anno fa, perché per ogni anno che passa l'aereo invecchia di più e vale di meno. Se non è stata venduta quando i velivoli avevano un anno di vita in meno, ci chiediamo oggi a quale valore possa essere venduta. Inoltre, essi ci dicono anche che l'Alitalia avrebbe una sua collocazione nel mercato internazionale, se avesse dei velivoli a lungo raggio

dei velivoli, secondo quanto emerso nell'indagine conoscitiva, sarebbe necessario un investimento di almeno un miliardo l'anno, per i prossimi anni. Chi ce lo mette questo miliardo l'anno, per i prossimi anni, per rinnovare un parco aereo che è fatto di velivoli vecchi,

- e pochi rispetto alla possibilità che una compagnia possa stare nel mercato? Dunque, mi chiedo: se il Governo efficiente non è riuscito a creare le condizioni perché, in questo anno, l'Alitalia fosse venduta ad un potenziale acquirente che garantisse il vettore nazionale in condizioni di mercato migliori dell'attuale, come può accadere questo nei prossimi mesi estivi?

in questi giorni la procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine per bancarotta fraudolenta nei confronti dei precedenti amministratori, Siamo preoccupati - e concludo - anche a fronte del fatto che il bilancio del 2016 non è stato ancora pubblicato,

emersi - di fatto, i conti sono già in condizioni tali da non poter restituire il prestito - sia per le condizioni della compagnia aerea, che ha una flotta sempre più antiquata, a fronte di un mercato del petrolio che oggi è ai massimi storici. Nel frattempo, però, per cercare di dare un indirizzo a chi verrà, abbiamo presentato e sono stati recepiti tre ordini del giorno, che hanno un loro preciso significato politico. L'ultimo lo ha esposto il senatore Fazzolari e riguarda il sistema aeroportuale,

due differimenti tecnici e altrettanto inevitabili, pesa il clima di incertezza politica e, anche se questa frase è stata cassata dal testo dell'ordine del giorno che noi del PD avevamo presentato, è un dato di fatto. È un fatto perché,

i nostri interventi in sede di Commissione speciale auspicando che un Governo, che in quel momento sembrava in predicato di poter essere costituito, potesse assumere decisioni importanti quanto gravi. Adesso ci siamo rituffati in un clima di enorme incertezza politica in cui, minuto dopo minuto, le cose cose evolvono e non sappiamo quale sarà il punto di arrivo. Quello di Alitalia è uno dei temi più gravi che avrebbero bisogno di governabilità; soprattutto di governabilità fatta in modo serio, con quella stessa serietà con la quale il Governo in carica - ancora per pochi giorni giorni - ha affrontato la questione. Con una metafora più che appropriata, ci è stato detto in Commissione speciale che, mentre discutiamo, rischia di esaurirsi il carburante. Proprio una metafora che è quasi realtà: se le decisioni non saranno prese in tempi brevi, ci ritroveremo in una situazione *ante* 2 maggio 2017, quando a un certo punto sembrava che gli aerei rimanessero a terra e non potessero più alzarsi in volo, facendo perdere quella fiducia che, com'è stato detto bene ieri dalla senatrice Malpezzi, è uno dei primi fondamenti quando si parla di aerei, di voli, di trasporti di questo tipo. Non mi soffermerò sulla storia degli ultimi anni; bisognerebbe tornare almeno al 2008, quando si individuò nella CAI la soluzione ai problemi di Alitalia: non andò bene. Nel 2014 sembrò che la soluzione offerta da Etihad fosse di assoluto prestigio e valore, anche per l'importanza che sul piano internazionale avevano quegli investitori. Purtroppo, anche in questo caso, le cose non sono andate bene. Il piano industriale fu bocciato nel 2017 perché il consiglio d'amministrazione riteneva vincolante che i lavoratori apprezzassero e approvassero quel piano. Non entro nel merito di quella decisione. Fatto sta che quella decisione ha determinato immediatamente dopo il passaggio all'amministrazione straordinaria. È in quel momento che entra in gioco il Governo, qui rappresentato per il MISE dal viceministro Bellanova, dal viceministro Morando e dal sottosegretario Amici. Un momento drammatico in cui, appunto, le prenotazioni venivano disdette, la gente non sapeva più se potesse fare il biglietto con Alitalia e c'erano in cassa soltanto 74 milioni di euro, con una debitoria di 3 miliardi di euro. Il Governo è intervenuto con un prestito di 600 milioni, necessari a evitare un'interruzione del servizio pubblico. È intervenuto nominando un collegio commissariale che, a parere del PD, ha svolto in maniera assolutamente positiva il suo compito. Il collega Urso si chiedeva perché non ha accettato le offerte che fino a ora sono arrivate: perché sono del tutto insoddisfacenti. Le prime sette offerte, quelle pervenute entro il 15 ottobre ottobre 2017, sarebbero state dannose per Alitalia e per il Paese. Sono stati riaperti i termini, ce ne sono tre oggi sul tavolo: Lufthansa, easyJet e Wizz Air. La migliore, che sembrerebbe essere quella di Lufthansa, comporterebbe però però il licenziamento di 2.000 operatori su 12.000 - non è quindi una scelta che si possa fare a cuor leggero - oltre a interventi su costi, destinazioni, dimensione societaria. Il decreto-legge in esame prevede due slittamenti di date: il differimento al 31 ottobre

le regole della vita e degli spostamenti per ciascuno di noi. Hanno messo in atto soluzioni manageriali dopo anni di inefficienza e la contrattazione dei costi operativi. A proposito di flotta, non è stato detto che, purtroppo, molti velivoli di Alitalia sono in *leasing* e che, addirittura, è stato possibile, attraverso la mera contrattazione, passare da costi di *leasing* di 850.000 Democratico, l'azienda ha la necessità di potenziare ancora le tratte a lungo raggio, attraverso aerei e flotta, e ha bisogno di migliorare lo sfruttamento di Linate. Nella scorsa legislatura un autorevolissimo esponente di Forza Italia, peraltro lombardo, ha sostenuto in Commissione che forse qualcuno dovrebbe fare autocritica sulla scelta di Malpensa, che non è stata proprio una scelta felicissima. Da Linate sono state abbandonate le tratte a lungo raggio, lasciando spazi alle società estere che fanno un servizio che l'Alitalia non fa più. Invece, Linate deve tornare

scenari *macro*, che sono le due possibili opzioni che hanno in questo momento il Paese e il Governo (quando ci sarà). La vendita a una compagnia straniera, tenendo conto che la migliore delle offerte arrivate, che ho descritto in poche parole, non è ritenuta soddisfacente. Oppure - ed è quello in cui il Partito Democratico spera e crede - il rilancio della compagnia attraverso nuovi investitori, in grado di perseguire gli obiettivi predetti in modo virtuoso, convinto e convincente. Investitori che non si può inventare né il Governo in carica né quello che verrà. Investitori le cui regole sono dettate dal mercato, cosa alla quale noi del Partito Democratico teniamo e non rinunciamo. a ulteriori misure di sostegno, cui non crediamo e che peraltro non sarebbero consentite dall'Unione europea. Colleghi, diciamoci con chiarezza che il terzo scenario sarebbe il *default* della compagnia. *Default* della compagnia significa perdere un gioiello del Paese. Rinunciare a una grande

terza drammatica opzione. Per questo ha lavorato il Governo, e bene. Per questo ha lavorato il collegio commissariale e per questo noi diamo un voto convinto all'approvazione del provvedimento. Speriamo che lo stesso senso di responsabilità, la stessa volontà di avere a cuore soprattutto i posti di lavoro dei nostri concittadini siano sentiti, percepiti e vissuti dagli altri partiti rappresentati in quest'Aula. *(Applausi

recante misure urgenti per assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. In particolare, il il termine per l'espletamento di tali procedure viene differito dal 30 aprile 2018 al 31 ottobre 2018, la durata del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro viene prorogata al 15 dicembre 2018. Il finanziamento viene incrementato di ulteriori

Ugo Arrigo e Gaetano Intrieri, entrambi favorevoli a un ritorno alla nazionalizzazione. Abbiamo sentito i commissari straordinari Gubitosi, Laghi e Paleari, il presidente di ENAC Riggio e il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione. Durante l'intera indagine conoscitiva, seguita da tutti i commissari con grandissima attenzione, è emerso un quadro di incredibile complessità, con la consapevolezza da parte di tutti che chi aveva la responsabilità della gestione nel passato ha portato a uno stato di insolvenza finanziaria e all'amministrazione straordinaria della società per delle scelte scellerate

Nell'ultima gestione con Etihad sono stati stipulati dei contratti incredibilmente svantaggiosi. Ciò ha provocato in tutti noi - si è sentito negli interventi in discussione generale uno stato di rabbia e frustrazione, perché tutti stiamo dicendo che Alitalia è la compagnia nazionale della quale dobbiamo essere orgogliosi per la qualità dei servizi, per la formazione del personale e dei piloti.

Sono stati sistematicamente stipulati dei contratti svantaggiosi per gli accordi sul carburante, per il noleggio degli aeromobili, per l'esternalizzazione delle manutenzioni, per il sistema dei costi di prenotazione dei biglietti e per i corsi del personale già formato fatti ad Abu Dhabi. E aggiungo la vendita di *slot* pregiati e i tagli di voli su rotte di lungo raggio.

Alcuni sindacati sostengono che c'è stato da parte dei lavoratori, con l'aumento della produttività e la riduzione degli stipendi, un finanziamento ipotetico di 700 milioni.

Quindi, si richiama il tema dello spezzettamento. Presenta effettivamente forse l'offerta più seria. Mette sul piano delle trattative 300 milioni, ma chiede garanzie sul risanamento e

una parte proveniente da Air Berlin, di cui Lufthansa ha acquistato il grosso degli *asset*. Non si capisce,

Nel 2017 ha già raggiunto 500 tratte e 144 destinazioni e ha come *hub* principale Budapest. Già da queste tre offerte più interessanti e serie si comprende come l'idea sia quella

della Lega voterà a favore di questo provvedimento per dare la possibilità di altri tre mesi per la ricerca di nuove offerte interessanti. Rimangono le considerazioni fatte dal collega Urso, che effettivamente le nuove contrattazioni avverranno in un periodo maggiormente sfavorevole rispetto a quello appena trascorso: il prezzo del carburante è salito

ritornando sulle tratte di lungo raggio, dove lo spazio è maggiore, dove le possibilità di sviluppo e di espansione sono notevoli e dove le qualità del nostro vettore nazionale potrebbero fare

una posizione dignitosa del nostro Paese. Lo vedremo nei mesi a venire e certamente sarà al centro dell'interesse del prossimo Governo che speriamo

il complesso aziendale che fa capo ad Alitalia SpA, è di fatto un provvedimento che sposta semplicemente la scadenza del 30 aprile 2018, quindi è una proroga

in questa sede questa mattina, che ha ricevuto il voto contrario da parte del nostro Gruppo. Si tratta dei primi due emendamenti votati da quest'Assemblea, che prevedono l'obbligo per i commissari di Alitalia di trasmettere alle Camere, ogni sessanta decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una relazione contenente informazioni puntuali. Il nostro voto contrario - che motivo in questa sede, anche se è già avvenuto - riguardava proprio gli obblighi eccessivamente stringenti: in fondo, i commissari Alitalia

troviamo all'interno di procedure che presentano elementi di riservatezza e sensibilità. In questa fase di valutazione, è emerso purtroppo anche il negativo risultato delle nozze con Etihad, che hanno impoverito la società di bandiera, con una riduzione della flotta e una tipologia di velivoli attualmente di difficile organizzazione, così com'è emerso

il rischio d'infrazione per la proroga del prestito, certamente, ma anche in questo caso credo debba esserci un confronto con l'Unione europea. L'interesse nazionale, in questo frangente, deve trovare una composizione con le regole dell'Unione europea, ma ricordiamo che il finanziamento da parte dello Stato non è di per sé stesso vietato da parte dell'Unione europea: deve avvenire a prezzo di mercato e, in questo caso, il prezzo di mercato, applicando una regola del 2008,

è comunque la compagnia che rappresenta un Paese (poi, la definizione giuridica di compagnia di bandiera è tutta un'altra questione). Alitalia ha abbandonato quasi totalmente il lungo raggio nel periodo di Etihad. Etihad. Negli ultimi anni prima dell'amministrazione straordinaria ha tenuto una strategia industriale esattamente opposta a ciò che avrebbe dovuto fare la compagnia di bandiera di un Paese come il nostro, che ha beni artistici e risorse culturali e turistiche (come hanno avuto modo di esprimere colleghi anche del mio Gruppo intervenuti) superiori al resto del mondo (messo tutto insieme il resto del mondo) al centro del Mediterraneo, con la possibilità di essere un grande *hub*. Purtroppo non è così: su 118 aerei solo 41 sono di proprietà.

esclusa da accordi fatti da altri gruppi. Con favore abbiamo appreso, invece, che grazie anche, in parte, agli accordi sindacali la questione, sollevata più volte, dell'eccedenza del personale, prevalentemente di terra, è in via di soluzione ancorché vi sia ancora una quota considerevole di cassa integrazione.

Colleghi, non è una questione di proprietà, non è il pur importante salvataggio di un'impresa, peraltro tutto pubblico, tutto privato o misto, con le valutazioni che si potrebbero fare: è una questione nazionale che pone alla nostra attenzione il quesito di quale percorso di sviluppo vogliamo intraprendere come Paese. Siamo un Paese che può essere una miniera per il turismo, che ha un terzo del prodotto interno lordo legato al rapporto con l'estero e che - ahimè - ha anche un terzo del debito pubblico legato all'estero, e in questi giorni ce ne stiamo Il non essere centrali nel settore del trasporto aereo è un danno collettivo, ecco perché Alitalia non è un'azienda qualsiasi. Il rischio di marginalizzazione quale periferia di Parigi o Francoforte è altissimo.

Se, con una compagnia in equilibrio, Fiumicino, Malpensa e Linate (che invece può fare tratte di lungo raggio e lo fa con altre compagnie) ridiventano un punto

i commissari siano accompagnati nei prossimi sei mesi nell'azione di risanamento e di rilancio intrapresa. Ci sia valutazione, si possano riacquistare gli *slot* ceduti e si trovi il *partner* finanziario o gestionale, come da mandato di legge. Onorevoli colleghi del Senato della Repubblica, una digressione mi sia permessa rispetto al tema specifico Alitalia: il presidente della Commissione speciale, senatore Vito Crimi (che ringrazio, unitamente al relatore), ha dichiarato inammissibili per materia - e io credo correttamente, perché ultronei rispetto alla materia

Non ha aperto il provvedimento, come suol dirsi, e non lo ha fatto diventare un treno. Credo tuttavia che, in questo difficile frangente,

debbano dare una risposta tempestiva anche ai temi contenuti in quegli emendamenti che avevano un'urgenza e che riguardavano gli investimenti sugli enti locali e la fatturazione elettronica. Nel merito, naturalmente, ogni forza politica ha la libertà di esprimersi, ma il Paese non può fermarsi. Forza Italia, con il senso di responsabilità che ci ha caratterizzati in questa fase e ci caratterizza nel difficile momento politico e istituzionale che stiamo vivendo, non viene meno al dovere di valutare nel merito e quindi voterà a favore di questo provvedimento. Signor Presidente, ci troviamo un'altra volta in quest'Aula a parlare di Alitalia, così come accadde nella scorsa legislatura e ci troviamo sempre a parlare di una compagnia in grande sofferenza.

dell'IRI. Con il primo Governo Prodi, nel grande periodo delle privatizzazioni, fu ceduto al mercato poco meno del 40 In quello stesso periodo, venne ceduta al mercato la gran parte di un'altra società pubblica: Telecom Italia. Nel 2000 il matrimonio di Alitalia con KLM fallì, perché KLM voleva che Malpensa fosse il centro delle operazioni, piuttosto che Fiumicino. L'anno prima, Telecom Italia era stata scalata a debito, scaricando il debito su Telecom. Mi pare che quell'operazione fu fatta da tale Roberto Colaninno.

mentre la trattativa era in corso, cambiò il Governo e arrivò il quarto Governo Berlusconi, che disse*: «*Alt! Non possiamo cedere la nostra compagnia ai francesi: facciamola tenere agli italiani». E arrivarono i capitani coraggiosi; fu creata una *bad company*, gli esuberi e il passivo furono posti nelle mani dello Stato e i capitani coraggiosi - che erano molto coraggiosi - presero in mano la compagnia.

(che potenza, questa famiglia!); poi c'erano Ligresti, Caltagirone, Tronchetti Provera. E chi diventa presidente di questa società? Sempre Roberto Colaninno, quello che aveva scalato Telecom a debito, il cui figlio, se non ricordo male, era il consigliere economico del Partito Democratico. Così mi sembra di ricordare, sono giusto sprazzi di memoria, così ricordiamo queste cose. Nel 2013 Alitalia è sull'orlo del fallimento, un'altra volta. Nel 2014 arriva il senatore semplice (così si è definito), il segretario del Partito Democratico,

si incrociano. Telecom era un'azienda *leader* in Europa, un'azienda che voleva realizzare il piano Socrate, che voleva portare, prima della privatizzazione, nel 1998, la fibra ottica a casa degli italiani,

che è sempre uno dei cosiddetti capitani coraggiosi: si incrociano sempre questi nomi, queste famiglie, queste situazioni,

la politica deve tutelare l'interesse collettivo, non l'interesse di questi signori. Ma evidentemente sia il Governo Berlusconi che quello del Partito Democratico hanno fatto esattamente il contrario di quello che era l'interesse collettivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ce lo dobbiamo ricordare, perché se non ricordiamo la storia, non andiamo da nessuna parte.

e si sono innamorati di questo capitale fluttuante, dove i cittadini non contano niente. Per non parlare dei lavoratori: se nel 2008 Alitalia aveva 23.000 dipendenti, siamo scesi, quando arrivò Etihad, a

Queste due storie si intrecciano profondamente, perché non c'è stata più una visione di questo Paese. Noi questo è ciò che avremmo voluto fare. Ma se non lo faremo oggi, lo faremo domani

fare! Voi vi siete persi, perché avete smesso di amare questo Paese. Sono chiacchiere quelle che dite quando dichiarate di amare questo Paese. Voi amate solo quelle piccole cose dietro le quali vi nascondete, come il potere, quella cosa così triste che vi ha fatto diventare delle persone grigie. Mi sembra che ne parlasse Gaber quando diceva che

Quando questa situazione finirà e non avremo un vuoto totale dove non c'è nessuno che può decidere, quando il Parlamento è sovrano e potrebbe indubbiamente decidere... ma con una situazione così con chi parliamo, se non c'è il Governo?

strane cose. Ad esempio, abbiamo letto che la procura di Civitavecchia sta indagando gli amministratori delegati del periodo Etihad, tra cui compare Montezemolo. Per carità, anche lui mi sembra che sia un nome noto: lo stesso Montezemolo che era socio di quell'Italo che ha venduto a 2 miliardi di euro, quando il capitale versato, cioè i soldi che hanno investito, era poco meno di 300 milioni di euro. Che cosa bella fare le plusvalenze!

cosa simpatica! Poi abbiamo parlato del fatto che non ci sono i dati. I dati sono qui. C'è una relazione pubblicata sul sito di Alitalia con la situazione patrimoniale. Nella situazione patrimoniale, aggiornata al 28 febbraio 2017, si scoprono delle cose interessanti, e cioè che Alitalia, dei 3 miliardi di indebitamento che aveva fatto per avere cassa, ha destinato 1 miliardo in strumenti finanziari, di cui 400 milioni in derivati e 600 milioni in crediti finanziari per pagare in anticipo le manutenzioni. È finanza, questa roba, o è un giochetto? Noi vorremmo capire chi paga. Perché se avete nominato come commissario straordinario anche una persona che si chiama Laghi, che era il capo del consiglio di amministrazione della Midco, che era l'azionista di maggioranza di CAI,

Allora, come si gestisce questa cosa? Si gestisce in un solo modo: mandando a casa chi è stato incapace, individuando le responsabilità, civili o penali; qualcuno deve pagare, ma non è possibile che continuino a pagare i cittadini italiani e i lavoratori. Questo è l'unico motivo per il quale noi siamo favorevoli a questa proroga, perché c'è bisogno di qualcuno che sappia pensare. Voi avete dimenticato il cervello a casa.

nuova finestra"). Onorevoli colleghi, come ricordato nella giornata di ieri dal presidente Casellati, è venuto a mancare Alberto Mieli, uno dei testimoni più attivi della tragedia dell'Olocausto. Desidero, anche a nome mio e di tutti i colleghi dell'Assemblea, esprimere ai familiari e all'intera comunità ebraica i sensi del mio profondo cordoglio e quello del Senato della Repubblica per la scomparsa di Alberto Mieli. Invito ora i colleghi a osservare un minuto di silenzio.

recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento in esame riguarda la conversione in legge del decreto-legge n. 30 del 2018, che reca norme dirette ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, mediante la proroga della durata in carica dei suoi componenti. È opportuno ricordare che l'Autorità di regolazione ARERA (ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) ha funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti. L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza; ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; a definire adeguati livelli di qualità dei servizi; a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. La legge 14 novembre 1995, n. 481, ha inizialmente individuato per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas competenze nei settori dell'energia elettrica e del gas. Le competenze regolatorie riconosciute dalla legge istitutiva in materia energetica sono state nel tempo ampliate e specificate, parallelamente all'evoluzione del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia a livello europeo. In particolare, in attuazione delle direttive del terzo pacchetto, il decreto legislativo n. 93 del 2011, successivamente modificato, ha specificato ulteriormente le funzioni dell'Autorità.

sono state trasferite all'AEEG le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già attribuite alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. I commi da 527 a 530 della legge di bilancio 2018, infine, hanno attribuito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. La normativa vigente, dunque, nel disciplinare l'istituzione dell'ARERA, quale organismo collegiale indipendente, prevede che i suoi cinque membri durino in carica sette anni e non possano essere confermati. La procedura, in particolare, dispone che essi siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, dopo l'acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'attuale collegio, nominato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2011, è giunto pertanto a scadenza lo scorso 11 febbraio. Dopo tale data, in forza di una deliberazione adottata l'8 febbraio 2018, l'ARERA ha continuato a operare in regime di specifica *prorogatio*, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del collegio, ed esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti; ciò in adesione al parere n. 5388 del 2010 espresso dal Consiglio di Stato proprio in relazione all'applicabilità dell'istituto della *prorogatio* al collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato degli attuali membri ha, quindi, reso necessaria l'adozione del provvedimento in esame, finalizzato a scongiurare l'interruzione delle attività a consentire che, alla nomina dei nuovi componenti, provveda il nuovo Governo. Il testo del decreto-legge si compone di due soli articoli. L'articolo 1, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli attuali componenti dell'ARERA continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018. Il testo originario del decreto fissava, quale termine per l'esercizio delle funzioni *in prorogatio*, il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Presso la Camera dei deputati è stato inoltre aggiunto un nuovo comma 1-*bis*, con il quale si prevede che, durante il periodo di *prorogatio*, l'ARERA trasmetta alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Il comma prevede inoltre che, nella prima relazione, l'Autorità dia conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili e urgenti. A tale ultimo riguardo occorre ricordare che nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione speciale della Camera, si è proceduto all'audizione, il 23 aprile 2018, dei rappresentanti dell'ARERA, i quali hanno segnalato, tra l'altro, di aver adottato preventivamente delle linee guida interne volte a individuare *ex ante* macro tipologie di atti qualificabili di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti. In tale ambito, sono stati ritenuti adottabili quegli atti che prevedano determinati presupposti preventivamente stabiliti dalle leggi nazionali, dalla normativa europea o da pregressi provvedimenti amministrativi. L'articolo 2 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In conclusione, vorrei ringraziare il funzionario della Commissione speciale, nella persona del dottor Alessandro Goracci, e tutti i suoi collaboratori per il supporto e il lavoro svolto nel corso dell'esame di questo decreto-legge,

Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore è stato esaustivo e ha già spiegato in maniera

Un primo nodo - li cito solamente, quasi per titoli, perché non è certamente questa la sede per un dibattito - è relativo alla determinazione delle tariffe efficaci che mirano, appunto, all'efficienza del sistema delle infrastrutture e delle reti. reti. È certamente questa una problematica di particolare rilevanza, rispetto alla quale si sono susseguite alcune sentenze di giudici amministrativi che hanno sancito il fatto che l'insoluto degli oneri elettrici vada pagato dai consumatori. Questi oneri sono stati generati da motivi diversi, quali la crisi di alcune società elettriche, errori di natura commerciale, condizioni di mercato, oppure dalla morosità di alcuni clienti.

È nostro parere che questo non debba avvenire, perché - e l'ultima legge di bilancio lo ha riconfermato - si è ritenuto che fosse un passaggio importante per garantire una qualità di servizi simile per tutta l'area del nostro Paese. A tal riguardo, è importante sottolineare che l'azione dell'Autorità dell'Autorità è diretta, per tutti i settori in oggetto di regolazione; a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza; ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizio in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; a definire adeguati livelli di qualità di servizio; a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefinibili, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Questa è la *ratio* - un criterio di omogeneità su tutto il territorio nazionale - che configura da parte nostra il mantenimento delle reti ambientali all'interno dell'ARERA stessa. Vi è poi un altro nodo importante che è il funzionamento e della relazione tra gli enti regolatori e gli enti regolati:

sto parlando del servizio idrico - che sono, in media nazionale, superiori al 30 per cento, ma addirittura superiori al 50 per cento in molte parti del nostro Paese. infine il tema del costo dell'energia elettrica per le famiglie in maggior tutela: sappiamo che alla fine di dicembre l'Autorità, nelle sue valutazioni, ha aumentato di circa

In principio l'Autorità aveva immaginato, con delibere *ad hoc*, la tutela da insolvenza di venditori e da qualsiasi altra situazione con polizze assicurative che avrebbero coperto queste evenienze. Il TAR ha pronunciato una sentenza avversa a questa lettura. Ora una revisione e un lavoro di raccordo sarebbero auspicabili per trovare una soluzione al problema. In ultimo vi è la questione relativa al *referendum* del giugno 2011

In realtà sulla vicenda si è già espressa la sentenza del Consiglio di Stato n. 2481 del 2017 intervenendo su sentenze del 2014 del TAR Lombardia sulla base di ricorsi fatti da alcune associazioni di consumatori, ricorda che il *referendum* che avrebbe obbligato l'affidamento del servizio idrico integrato esclusivamente ad aziende di diritto pubblico in realtà non si è mai svolto. infatti, di un *referendum* che non passò il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale e, quindi, non passò mai sotto la penna del popolo sovrano. Il *referendum* che invece arrivò alla matita del popolo, assieme a quello che cancellava l'obbligatorietà della gara o della concessione del 40 per cento del capitale per i servizi pubblici a rilevanza economica, era quello che aboliva, nella voce di formazione della tariffa idrica, la remunerazione forfettaria, che all'epoca era fissata al 7

che tale remunerazione fosse calcolata ispirandosi al principio del *full recovery cost*. In sostanza, il principio stabilito dalla sentenza invece, veniva contestato dai presentatori del ricorso al TAR - è che nel caso in cui siamo effettivamente in presenza di investimenti, attingendo sia al credito privato che alle risorse proprie dell'ente, venga riconosciuta la tariffa sul costo pieno, mentre i sostenitori del ricorso negavano la possibilità nel caso in cui si attingesse alle risorse proprie dell'ente.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge in discussione ha un valore squisitamente tecnico e per questa ragione il nostro Gruppo non ha particolari osservazioni da fare. Reputiamo di buon senso il fatto che l'Autorità, in fase cautelativa, abbia adottato delle linee guida per stabilire gli ambiti di intervento di ordinaria amministrazione

le Aule del Parlamento dovranno tornare a occuparsi di ARERA prima del 30 settembre, quando scadrà la proroga che stiamo votando. Da questo punto di vista ARERA è solo un esempio di quello che succede a causa di un prolungato periodo di incertezza politica. Crediamo ci sia materia su cui riflettere, così come ce n'è stata per Alitalia, per tutte quelle urgenze e problemi che richiedono una stabilità della politica e delle istituzioni. Gli ambiti di intervento dell'Agenzia sono tanti e tutti di straordinaria importanza: non solo l'acqua o l'energia, ma anche il tema importantissimo del conferimento dei rifiuti. Su questo, in Commissione, è stato presentato un ordine del giorno e il Governo, giustamente, si è esentato dall'assumere impegni, ribadendo che è in carica per gli affari correnti. In ogni caso, il mio auspicio è che i parlamentari di questa o della prossima legislatura tengano in doverosa considerazione tutti questi temi, che sono strategici e riguardano i consumatori e in qualche modo anche i diritti di cittadinanza, se si pensa a quelli dell'acqua o della cura dell'ambiente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si rende necessario a seguito della scadenza, avvenuta lo scorso 11 febbraio, del collegio dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva dell'Autorità, la legge n. 481 del 1995, la durata dei componenti e del Presidente del collegio è di sette anni non rinnovabili. Il fatto che il termine del mandato coincidesse con la scadenza naturale della legislatura ha portato il Governo Gentiloni a non procedere con la nomina e la formazione del nuovo collegio, per rispetto istituzionale verso il nuovo Parlamento. dunque - come è desumibile da apposito parere del Consiglio di Stato - lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità, seppur ridotte agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili e urgenti, è proseguito in regime di *prorogatio*. In forza di una deliberazione adottata l'8 febbraio 2018, l'ARERA ha continuato a operare in regime di specifica *prorogatio*. Tuttavia, la *prorogatio* non può eccedere i sessanta giorni come da parere del giudice amministrativo e, pertanto, l'11 aprile 2018 il regime si è concluso. L'ulteriore prorogabilità avrebbe potuto configurarsi solo con un'apposita disposizione normativa e da qui nasce la necessità di un decreto-legge come quello al nostro esame, finalizzato a consentire a un'Autorità di svolgere funzioni davvero fondamentali, vale a dire la regolamentazione di settori industriali chiamati ad assicurare la fruizione di servizi pubblici di primaria utilità. Durante l'esame del provvedimento presso la Camera sono state introdotte due modifiche molto importanti e condivisibili: la prima riguarda la definitiva chiusura del regime di *prorogatio*, fissata inderogabilmente al 30 settembre; settembre; tempi certi che in un contesto politico ancora caratterizzato da elevatissime incertezze offrono però una scansione temporale in grado di consentire la formazione e, quindi, la piena operatività la piena operatività di un'Autorità così importante per la gestione dei sistemi energetici, idrici e ambientali. La seconda modifica consiste nell'assicurare al Parlamento il controllo sulla natura dell'ordinaria amministrazione e dell'indifferibilità e dell'urgenza degli atti attraverso la trasmissione alle Camere, ogni quarantacinque giorni, di una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione. Il ruolo del Parlamento acquisisce la dovuta centralità, anche in merito alla procedura di nomina dei nuovi componenti.

esso stabilisce altresì che le designazioni del Governo debbano essere sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e in nessun caso le nomine possano essere effettuate in mancanza di parere favorevole espresso dalle suddette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Si tratta, dunque, di un provvedimento complesso e particolarmente rafforzato, nel quale il ruolo del Parlamento non è irrilevante e, data la presenza di un *quorum* qualificato e alto per la scelta dei componenti dell'Autorità, contribuisce a garantire la necessaria professionalità e competenza nella regolamentazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità quali l'energia, le risorse idriche e l'ambiente. Nei principali settori di monopolio naturale - energia elettrica, risorse idriche e ciclo dei rifiuti - abbiamo un soggetto regolatore molto grande. Vale la pena ricordare che l'Agenzia ha visto crescere progressivamente le proprie competenze. Nasce, infatti, in un primo momento come Autorità per l'energia elettrica e il gas; successivamente con decreto n. 201 del 2011 (il cosiddetto decreto Salva Italia) ha acquisito competenze sul settore idrico e infine, con l'ultima legge di bilancio, ha assunto la competenza anche nel settore del servizio integrato dei rifiuti. Se qualche rilievo è consentito, al fine di stimolare una futura discussione e sperabilmente di contribuire a rendere maggiormente efficace ed efficiente la regolamentazione nella prospettiva di un servizio sempre più adeguato e con costi per consumatori e utenti più ridotti, una prima considerazione non può che riguardare la discrasia rispetto al ruolo che l'Agenzia svolge con riferimento ai settori del gas ed elettricità, da una parte, e dell'acqua e dei rifiuti, dall'altra. Relativamente ai primi due settori, l'Autorità stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, mentre per gli ultimi due settori la competenza della suddetta Autorità riguarda la determinazione la determinazione del metodo tariffario e dell'approccio alle tariffe, che sono invece determinate da altri soggetti, ovvero dalle Autorità di ambito territoriali. Si pone, allora, un problema che dovremmo iniziare ad affrontare, se vogliamo che la gestione di determinati servizi possa svilupparsi meglio e in termini di efficienza e di contenimento dei costi per l'utenza. Un primo problema riguarda l'asimmetria dimensionale tra il soggetto gestore delle risorse idriche - ad esempio - e il soggetto regolatore, le Autorità d'ambito, laddove queste ultime hanno una dimensione provinciale o, al massimo, regionale, mentre non sono rari i casi di soggetti gestori di dimensione sovraregionale, addirittura quotati Il regolatore arriva molto spesso con molta difficoltà e anche con ritardi a conoscere esattamente i costi effettivi dell'affidatario del servizio, e ciò aumenta i problemi in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio. Se quanto detto è vero, lascio al futuro dibattito il tema di come affrontare il ruolo dell'Agenzia quale soggetto preposto allo svolgimento di un ruolo ancora più incisivo nella determinazione tariffaria.

che non raramente assommano il ruolo di gestori (presenza dei sindaci negli ambiti territoriali) e di affidatari del servizio di pubblica utilità (presenza del Comune nel capitale sociale dell'impresa affidataria). Come può un sindaco essere soggetto regolatore e soggetto regolato al tempo stesso e garantire una piena concorrenzialità del mercato, attraverso la scelta dell'operatore più efficiente, se l'amministrazione che è chiamato a guidare come sindaco figura come socio o come proprietario di una delle imprese concorrenti? E ancora: come può regolamentare un servizio raggiungendo livelli ottimali di efficienza e di riduzione dei costi per gli utenti, quando l'essere socio o proprietario dell'impresa affidataria determina entrate consistenti in grado di meglio garantire gli equilibri economico-finanziari del Comune che egli stesso amministra? Ecco, riflettere sulle criticità, alcune delle quali sono quelle appena ricordate, riguardanti la gestione dei servizi di monopolio naturale e di pubblica utilità potrebbe aiutare a ottenere un'erogazione di servizi ai cittadini sempre più ottimale in termini di efficacia, di efficienza e di costi. *(Applausi

Signor Presidente, gentili colleghi, da parte del Gruppo Forza Italia assicuro il voto favorevole: ci pare un atto dovuto di fronte al lavoro della Commissione speciale e della Camera. Sono state ben spiegate le modifiche che la Camera ha apportato, sulle quali concordiamo, perché la fissazione di un termine di novanta giorni dal giuramento del primo Governo

spiegati dal relatore, poiché questa negli anni ha cambiato nome avendo assunto nuove competenze: si tratta delle funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti. È un settore immenso - manca solo la telefonia,

del patrimonio infrastrutturale che porta i servizi è, infatti, un valore assoluto per il Paese, anche perché offre dei vantaggi in termini di economicità e probabilmente anche di risparmio per gli utenti. Ci piace pure che la legge di istituzione dell'Autorità abbia previsto - come è capitato per altre *Authority* - che i membri del collegio non possano essere riconfermati dopo i sette anni

- non è possibile - possa discutere prossimamente di alcune cose che vado rapidamente a elencare e che obbediscono ad alcuni princìpi che credo possano essere condivisi. Noi dobbiamo sempre mirare alla sostanza dei problemi e non alla forma.

faccia sì che i contratti *standard* per la fornitura dei servizi siano chiari, scritti in caratteri leggibili, non vessatori; anche se sappiamo che, a seguito di disposizioni di legge, tutte le clausole che possono avere una venatura di danno rispetto all'utente devono essere controfirmate. Ma la mia affermazione rispetto a certi contratti credo possa sussistere. Penso che ARERA debba controllare i gestori, anche perché a volte l'attuazione delle norme è più lenta di quanto pensiamo e possono esserci anche delle violazioni, perlomeno minimali. A tale proposito, ritengo debba essere vigilata l'attuazione della norma che prevede il divieto dei maxiconguagli, anche al fine di non mettere in difficoltà le famiglie. famiglie. L'Autorità deve educare al risparmio energetico personale e di sistema, anche se in questo c'è una contraddizione. Conosco un consorzio di rifiuti

In senso lato, il risparmio energetico o il risparmio su tutto questo sistema è una questione educativa molto importante. Penso debbano essere contenute le spese fisse in bolletta, perché queste ultime continuano a essere

Chi ripiana? I Comuni che sono soci? E per le società miste può valere lo stesso problema; le società private riescono più o meno a sopravvivere. Ma abbiamo uno stato di fatto, come si usa dire adesso, che riguardo al sistema elettrico è da terzo mondo. Ci sono dei pali che portano l'energia, soprattutto nelle zone di campagna, che toccano terra. Chi è amministratore locale sa che, se deve trattare con l'ENEL o con qualche altra autorità competente per far raddrizzare un palo, fatica e non poco. Il gas è un servizio più recente, le cui linee sono più o meno a posto, salvo il completamento e salvo le grandi linee internazionali. Non parliamo del sistema dell'acqua, dove le condutture in certe zone sono un colabrodo e dove le fognature sono un *optional* o dei rifiuti, con le discariche e gli impianti di preselezione (lo vediamo in tante situazioni). In conclusione, c'è una necessità di investire cifre macroscopiche, miliardarie. Qualcuno aveva ipotizzato che si facesse fronte

pubblica che finanzi gli investimenti affinché l'economia si rimetta in moto e affinché dagli investimenti derivino nuove entrate - come prevedibile - e si risolva in parte anche il problema dell'occupazione. perdoni, Presidente, se ho fatto questi accenni, ma credo che siano nell'ambito del discrezionale, degli auspici a quest'Assemblea per il futuro, augurandoci di poterne discutere pacatamente.

è molto complesso e richiederebbe sicuramente un'analisi più accurata, ma al di là dell'immediata contingenza delle scadenze, credo che questa discussione generale possa permetterci di evidenziare come questo decreto-legge presenti evidenti carenze. Ad esempio, c'è poco o nulla sulla proroga di graduatorie per l'assunzione di personale. Era doveroso, forse, in questa sede, rivedere anche la proroga per il personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l'ARERA. Così come poco è stato trattato l'impegno relativo al trasferimento delle competenze dell'ARERA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. impegno si pone peraltro in netto contrasto con quanto scritto all'interno del testo del provvedimento stesso. Infatti, ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del Regolamento, gli ordini del giorno devono recare istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Va quindi ben chiarito questo punto. Nel corso della sua attività, l'ARERA ha senza dubbio avuto il merito di razionalizzare il settore delle regolamentazioni, arrivando ad assorbire compiti e funzioni propri di altri istituti, fino ad arrivare ad inglobare, nel gennaio 2018, anche quelli relativi al settore dei rifiuti. Sembra che nel tempo l'azione dell'ARERA sia stata più aderente a criteri di mera economicità e di rappresentanza delle società responsabili del servizio che,

le sofferenze dovute alle morosità sulle bollette degli utenti virtuosi relativamente agli oneri di sistema non pagati dagli operatori e distributori di energia. Ciò è avvenuto anche nel campo dei rifiuti, con il recentissimo caso Umbria, che ricalca a pieno la precedente problematica. Ha fatto molto discutere, infatti, a ben vedere, la decisione dell'Autorità di addebitare ai consumatori 200 milioni di euro di bollette non pagate,

un termovalorizzatore che era stato previsto in un fazzoletto di terra nella zona della piana fiorentina, fortemente voluto dal PD locale e regionale insieme alla realizzazione

Casi analoghi, quindi, si stanno verificando in tutta Italia. Non possono essere i consumatori a pagare il danno che le società subiranno dai "buchi" derivanti dalla morosità di certi utenti o per errori di progettualità politica. È assurdo! È soprattutto però nel campo delle fruizioni dei servizi idrici che tali criticità sono emerse in modo chiaro, stante una pronuncia referendaria che, in molti casi, è stata in realtà disattesa proprio nel rapporto privilegiato tra l'ARERA e le società che gestiscono i servizi stessi. Ecco alcuni esempi: si è permesso che le difficoltà economiche di queste società consentissero l'applicazione di aliquote tariffarie in deroga, oppure che alcune delle società in oggetto continuassero in effetti a essere *borderline* rispetto al quesito referendario, essendo partecipate anche da capitali privati o comunque operanti con istituti di natura civilistica fossero applicate in bolletta voci, quali quelle relative al costo della risorsa finanziaria, che appaiono incompatibili con l'esito referendario o con l'applicazione di conguagli pesantemente retroattivi. quindi necessario riconsiderare alcuni aspetti della gestione dell'Autorità, valutando l'introduzione, pur nel rispetto dell'autonomia anche manageriale dell'istituto, di meccanismi che mettano l'Esecutivo e il Parlamento nelle condizioni di fornire le linee di indirizzo politico in base alle quali il collegio

opportuno introdurre verifiche periodiche, attraverso audizioni da tenere nelle Commissioni competenti, in merito all'operatività concreta della stessa e al campo delle proprie competenze. Gruppo Fratelli d'Italia ci chiediamo se la politica possa non considerare che gli aumenti generalizzati dei costi delle utenze rappresentano per le famiglie una voce di spesa sempre meno sostenibile e non prevedere, quantomeno, un un regime di controlli più serrati su tariffari e le rateizzazioni, in virtù dell'interesse generale. Riteniamo che, per questioni di indirizzo politico, il mero strumento legislativo, a fronte della quotidiana *governance* di tali settori, risulti comunque meno efficace se non affiancato, affiancato, appunto, da una costante opera di indirizzo e controllo che le istituzioni parlamentari dovrebbero essere in grado di effettuare. Proprio per i motivi suddetti Fratelli d'Italia ritiene che l'attuale discussione generale dovrebbe essere l'occasione per fornire analisi e proposte in merito.

Questo considerando alcune evidenti criticità contenute nel disegno di legge stesso, che derivano proprio dalle motivazioni portate a supporto dello stesso e contenute nella relazione tecnica. In buona sostanza, sia la legge costitutiva delle Autorità sia un parere del Consiglio di Stato, che una sentenza della Corte costituzionale sanciscono che una *prorogatio* dei membri dei collegi delle Autorità, per essere legittima e compatibile con la normativa vigente, deve rispondere fondamentalmente a due requisiti: essere di ragionevole durata e comunque non eccedere i sessanta prevedere che in regime di *prorogatio* l'attività dei collegi sia limitata all'ordinaria amministrazione. Nel disegno di legge si ipotizza, invece, una proroga *contra legem* a tutti gli effetti. Il collegio di ARERA, difatti, è scaduto l'11 febbraio 2018 e con la previsione di una proroga fino al 30 settembre verrebbe di fatto a essere prorogato per ben più di sette mesi. Fratelli d'Italia pensiamo che una proroga così ampia non abbia alcun senso e crediamo sia necessario fissare la proroga in trenta giorni, come previsto dall'emendamento presentato alla Camera dei deputati, che non abbiamo riproposto al Senato in quanto ritenevamo che in un Paese normale, con una maggioranza parlamentare conclamata, ad oggi avremmo potuto con un Governo legittimamente insediato, che avrebbe di fatto reso inutile la proroga. Concludo ponendomi e ponendo a tutti i colleghi una domanda. Oggi in Aula abbiamo affrontato due provvedimenti decisamente importanti per gli italiani. Il primo riguarda Alitalia, la nostra compagnia di la nostra compagnia di bandiera, e il secondo appunto ARERA, l'autorità regolamentatrice; due provvedimenti che influiscono e incidono in maniera tangibile sulle tasche dei cittadini. Il decreto-legge sull'Alitalia rappresenta la nostra finestra sul mondo;

avrebbero bisogno di essere ridiscussi in modo più approfondito ed esaminati nel dettaglio, ma l'attenzione al momento è molto più incentrata sulla situazione politica e istituzionale. Mi sorge quindi un dubbio e mi chiedo se i provvedimenti in esame siano stati inseriti volontariamente dal precedente Governo in questa fase, a causa dell'incapacità dello stesso di affrontare queste

Signor Presidente, il decreto-legge in esame detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prorogando la durata in carica dei rispettivi componenti. Il disegno di legge si compone di due articoli. In particolare l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione speciale esame atti di Governo della Camera con l'approvazione di un emendamento a firma del relatore, onorevole Dario Galli, dispone che i componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta autorità. Si specifica quindi il termine ultimo e inderogabile per l'esercizio di tali funzioni, individuato non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e comunque non oltre il 30 settembre 2018. Il testo originario dell'articolo prevedeva, quale termine per l'esercizio delle funzioni in *prorogatio*, il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nel corso dell'esame nella Commissione speciale della Camera è stato inoltre introdotto all'articolo 1 il nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che l'ARERA, durante il periodo di *prorogatio*, trasmetta alle Camere ogni una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento. L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno stesso della pubblicazione del decreto-legge Dopo l'esame della Camera, che ha introdotto alcune modifiche al testo (come dicevamo), il Senato ha solamente accolto due ordini del giorno durante l'esame presso la nostra Commissione speciale. Il decreto-legge alla nostra attenzione costituisce quindi quello che si può definire un atto dovuto per consentire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di continuare nelle proprie funzioni, prorogando la durata in carica dei componenti. I componenti dell'ARERA continueranno conseguentemente ad esercitare le proprie funzioni, ma limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Sono inoltre fissati limiti ben temporali ben precisi.

il buon funzionamento dell'Autorità, perché, considerati i tempi necessari per formare un nuovo Governo, stabilire un termine al 30 settembre potrebbe significare tranciare l'operatività dell'Autorità o almeno quella dei suoi componenti. Forse sarebbe stato più opportuno lasciare il termine dei novanta giorni, come previsto nel testo del decreto-legge: non abbiamo dubbi che il 30 settembre 2018 possa essere una data che rischia di necessitare un ulteriore decreto-legge di proroga. L'altra modifica introdotta dalla Camera è quella che riguarda la relazione alle Camere sull'attività svolta dall'Autorità. Una relazione ormai si chiede si chiede a tutti su tutto e non si nega a nessuno. Sarebbe utile, a questo punto, verificare chi le legge poi tutte queste relazioni, che ormai inseriamo in ogni provvedimento; non vorremmo che finissero solo per essere messe agli atti. Tra l'altro, per chi volesse documentarsi ulteriormente, va detto che l'Autorità ha un sito ricchissimo di determinazioni e di delibere da leggere e consultare. Ricordiamo solamente che i componenti dell'ARERA sono stati nominati nel 2011 e che la loro scadenza era appunto prevista nel febbraio 2018. Ricordiamo che la procedura di nomina prevede il parere vincolante, a maggioranza dei due terzi dei componenti, delle Commissioni parlamentari competenti sui nomi proposti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, approvati dal Consiglio dei Ministri. Questa procedura garantisce certamente un *quorum* di gradimento parlamentare molto alto, che di fatto comprende quasi tutte le forze parlamentari. Vanno ricordati al riguardo alcuni punti: che le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono dal bilancio dello Stato, ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati. La stessa Autorità ha volontariamente ridotto il contributo, che per legge è previsto all'uno per mille dei ricavi degli operatori, con differenziazioni in funzione del settore dell'attività svolta dai diversi soggetti: quindi, questo quadro rafforza la circostanza che l'Autorità possa operare in autonomia e con indipendenza di giudizio. Ovviamente il contesto in cui opera l'ARERA deve seguire gli indirizzi di politica generale del Governo e del Parlamento oltre che delle normative dell'Unione europea. ricordiamo che l'Agenzia opera in regime di *prorogatio*, che il Consiglio di Stato ha voluto limitare a sessanta giorni, prevedendo che in regime di *prorogatio* eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli che siano ritenuti indifferibili e urgenti. Quindi il decreto-legge era necessario a prorogare questo regime, che serve appunto a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorità. e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale: i servizi essenziali per i cittadini, quali l'energia elettrica e il gas, ma anche i servizi per l'ambiente. dalle decisioni dell'Autorità dipendono anche le tariffe a carico degli utenti, quindi essa ha compiti anche e soprattutto di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. È questo a nostro avviso il ruolo certamente prioritario dell'Autorità, quello di tutelare gli interessi dei consumatori attraverso l'attività di regolazione e di controllo delle tariffe, che riguardano i settori dell'energia e del gas. siamo accorti del nuovo quadro di regolamentazione del settore dell'energia dopo le telefonate che abbiamo ricevuto per passare a nuovi gestori nel mercato libero dell'energia. Quello che auspichiamo adesso, in maniera sempre crescente, è che possa emergere da questo mondo, da questo ambiente concorrenziale, una serie di tariffe migliori per l'utente finale, per i cittadini, soprattutto in settori come quello dell'energia, dove tutto sommato un certo livello di concorrenza negli ultimi anni è stato certamente innescato dalla normativa già adottata dal Parlamento. Concludo parlando del settore della gestione dei rifiuti, che pure interessa uno degli ordini del giorno al nostro esame, approvato dalla Commissione speciale, G1.100. Va detto che il Parlamento dovrà affrontare al più presto e in maniera coerente la complessa tematica della TARI, la tassa sui rifiuti. Non si può non notare che, dopo il blocco dell'aumento delle imposte locali, deciso dalle ultime manovre di bilancio, questa tassa sia diventata praticamente l'unica leva fiscale che hanno a disposizione i Comuni. Noi però riteniamo che questa tassa non possa concretizzarsi e affermarsi come una sorta di patrimoniale sulla casa, in cui il servizio reso dai gestori dei servizi ambientali non corrisponde, tra l'altro, nemmeno lontanamente alla tassa pagata. Auspichiamo quindi che il Parlamento possa certamente e prontamente porre mano a questa autentica ingiustizia, che va a penalizzare in modo subdolo il settore immobiliare, già fortemente danneggiato da una tassazione quasi quadruplicata dell'ultimo Governo eletto degli italiani, quello del presidente Berlusconi. Con questo confermo che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della proroga prevista dal decreto-legge

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in tutti gli interventi è stato sottolineato come, a prescindere dall'oggetto specifico del decreto-legge, la discussione generale sia l'occasione per richiamare l'attenzione del futuro Governo e del Parlamento sulla necessità di approfondire e rivedere le funzioni complessivamente attribuite all'ARERA. Non è un caso che questa richiesta sia corale, se si considera che appena il 27 dicembre 2017 sono state attribuite tali funzioni all'Autorità e che, allo stesso tempo, appena ad aprile scorso, il TAR del Lazio ha riconosciuto in materia di rifiuti la fondatezza del ricorso presentato in merito alla legittimità di parte dello sblocca Italia, in particolare relativamente Questo sottolinea come il tema dei rifiuti sia centrale e come il nostro Paese non possa limitarsi ad assegnare in maniera tecnica e formale all'ARERA una funzione di controllo e gestione senza approfondire il tema e in particolare, come indica anche l'ordine del giorno che la Commissione sottoporrà tra poco all'Assemblea, senza eliminare i contrasti tra le funzioni attribuite alle Regioni e quelle attribuite all'Autorità. Al Paese non serve un commissariamento delle Regioni virtuose, ma piuttosto

Signor Presidente, colleghe e colleghi, parliamo oggi di un altro argomento importante, al pari di quello che è stato discusso ieri e stamattina. stamattina. Lo stiamo discutendo e vivendo con lo stesso clima di ieri, con le stesse sensazioni e più o meno tutti con lo stesso atteggiamento, anche a giudicare da molte delle parole che sono state dette da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Nota dolente, il fatto che molto probabilmente servirà una nuova proroga, visto che la scadenza è prevista proprio in un mese fatidico, che sarà il prossimo settembre.

ma soprattutto - leggiamo nei suoi principi costitutivi - come ente indipendente. Questo è il punto centrale, secondo me,

evidenziato, se non addirittura denunciato, molti aspetti, alcuni dei quali sono stati già rilevati anche nel corso di questa discussione generale. Voglio aggiungere alcuni elementi che saranno importanti proprio in fase di proroga.

l'indirizzo fornito dalle Assemblee parlamentari, e questo ci suona come comune a molte altre denunce che abbiamo fatto in queste Aule. Non da ultimo il fatto che, in regime di *prorogatio*, l'Autorità ha emanato circa 188 delibere:

andando a scorrere i temi toccati da quelle delibere, non si capisce proprio perché queste siano state fatte in regime di *prorogatio*, dato che non vi era

al di là della sua competenza, a mio modo di vedere, e quindi andando a sconfinare in un campo che era molto più politico, piuttosto che di garanzia e di tutela. In molti casi, purtroppo, anche in questo settore e anche per questa Autorità abbiamo parlato di un Parlamento che è stato un po' esautorato dal suo potere di controllo. Purtroppo, questo è stato un po' il tema ricorrente della scorsa legislatura e, come stiamo vedendo anche in queste ore, è il tema ricorrente anche di questi pochi atti che stiamo discutendo.

per non cadere in questa proroga. Ma tant'è, siamo arrivati a questo punto. È chiaro che occorrerà un'attenta vigilanza nei prossimi mesi e nei prossimi anni, comunque sia,

dei temi toccati dall'Autorità è proprio l'acqua e - guarda caso - l'acqua è ancora, a tutti gli effetti, il primo punto che abbiamo scritto nel nostro contratto di Governo. L'acqua pubblica, l'Autorità garantisce proprio questo servizio. Noi abbiamo scritto in quel documento che l'acqua deve essere pubblica e che va tutelato il bene comune acqua, tra l'altro come volontà espressa con il *referendum* del 2011. Guarda un po': un altro tema di mancanza di tutela della sovranità popolare. Abbiamo parlato in quel documento della fondamentale importanza di ristrutturare la rete idrica, anche per rilevanti aspetti sanitari. Questo per poter fornire un servizio di qualità ai cittadini, a partire proprio dal bene fondamentale, dal bene comune acqua e, quindi, dalla qualità dell'acqua. Si tratta, quindi, di un argomento di rilevanza fondamentale, sul quale, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, il Parlamento dovrà essere attento sia con un'azione di controllo, ma soprattutto con una attenta guida politica. E che questa guida politica rimanga esclusivamente di controllo parlamentare. Concludo questo mio intervento semplicemente rivendicando il fatto che questa Autorità dovrà, sia durante questa proroga ma anche successivamente, avere un ruolo molto meno politico e più di garanzia per i servizi e soprattutto per i diritti dei cittadini.

dell'energia elettrica, del gas, dei rifiuti e dell'acqua; temi che, in un certo senso, hanno aperto un dibattito che mi auguro

finanze*. Signor Presidente, non intendo replicare. Vorrei solo dire che il dibattito si è concentrato sulle iniziative che, a questo proposito, si dovranno sviluppare nel prossimo futuro, con particolare riferimento a modifiche legislative. È noto che questo Governo è in carica per l'esercizio dell'attività di amministrazione degli affari correnti e non è in grado, secondo Costituzione, di sviluppare iniziativa legislativa. Signor Presidente,

l'opportunità di intervenire in questo settore, che riguarda gli utenti morosi, è un impegno che deve assumere il prossimo Governo. Il parere del relatore è ovviamente favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Al contrario, sarò costretto - l'ho detto all'inizio della precedente legislatura, quando il Regolamento era leggermente diverso - di volta in volta a chiedere sempre il voto elettronico. Credo che questa *impasse* potremmo superarla con un'interpretazione da parte

della seduta e non subito prima delle votazioni, come ben scritto Signor Presidente, avendo scritto anch'io la riforma del Regolamento, le sottolineo, al fine di velocizzare, che non c'è alcun ulteriore ragionamento rispetto a quello che le sto chiedendo. Suggerirei di utilizzare un pizzico di buonsenso nel consentire sempre di votare all'Aula con il sistema elettronico, che consente a tutti di potere votare in maniera veloce,

Si tratta, come nel caso di Alitalia, di un voto tecnico per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per gli atti di ordinaria amministrazione. Come già sottolineato in discussione generale, bene ha fatto l'Autorità ad adottare preventivamente le linea guida volte a stabilire le macrotipologie di atti indifferibili e urgenti e bene ha fatto la Camera a introdurre il comma con il quale si prevede che ARERA, durante il periodo di *prorogatio*, trasmetta ogni quarantacinque giorni una relazione riguardante gli atti che sono stati adottati. È giusto aver introdotto questi accorgimenti cautelativi in un'ottica di garanzia dei commissari e naturalmente dell'Autorità. Tuttavia, non dimentichiamoci che un'Autorità così importante, che riguarda settori di notevole rilevanza strategica, oggi non è nelle condizioni di operare pienamente. Non è un caso che in Commissione, rispetto all'ordine del giorno con cui si chiedeva di avviare una riflessione sui compiti e le funzioni di ARERA, il Governo abbia precisato di non poter assumere impegni che eccedano dall'ordinaria amministrazione. Per questo diciamo nuovamente che il nostro auspicio è che questa fase d'incertezza e instabilità si chiuda quanto prima: lo stallo dura da troppo tempo. Il Paese necessita di risposte e di un Governo che, in tutte le sue articolazioni e in tutti i suoi uffici, sia nella possibilità di fornire elementi di indirizzo.

competenti, sull'autoproduzione energetica e sulla questione dello scambio *in loco*. Pertanto, dal nostro punto di vista l'Autorità non ha svolto quel ruolo di avanguardia e di stimolo, non solo di mera regolazione e anche di garanzia della concorrenza in questo settore,

Non è un caso che, in particolare sul settore idrico, l'ARERA abbia svolto un ruolo a nostro avviso assolutamente negativo

non era certamente investita del potere di interpretare l'esito referendario, non ha eliminato la tariffa in qualsiasi modo riconducibile alla remunerazione del capitale investito. Questo è un tema che

il secondo provvedimento di questa legislatura, il secondo di questa giornata, il secondo provvedimento di proroga cui i Gruppi parlamentari si adeguano

e su questo noi ci pronunceremo come ci siamo pronunciati relativamente al decreto di proroga del commissariamento del prestito dell'Alitalia, anche in quel caso un decreto e una proroga politica. In quel caso però ci siamo astenuti astenuti per non creare ulteriore allarme e preoccupazione nel comparto e soprattutto tra i lavoratori che sono impegnati, giustamente, a difendere e a tutelare il vettore nazionale. In questo caso invece il nostro voto, come alla Camera, sarà contrario. Sarà contrario in termini di diritto. Voglio far notare ai colleghi parlamentari che questa *Authority* ha una vita di sette anni. Quando fu nominata, ormai ben più di sette anni fa, il contesto era del tutto diverso, era un'*Authority* per l'energia e il gas. Nel frattempo ha assunto ulteriori competenze, l'ultima delle quali con l'ultima legge di bilancio, particolarmente importante perché riguarda il ciclo dei rifiuti. Quando i commissari furono scelti, evidentemente lo furono per le loro competenze sull'energia e sul gas. Credo non abbiano le stesse competenze sul ciclo dei rifiuti o sui problemi idrici, quindi emerge macroscopicamente un problema di inadeguatezza.

peraltro con una proroga legislativa a fronte di una proroga già fatta su un parere del Consiglio di Stato dalla stessa *Authority*, che si è autorigenerata.

tra poche ore) ancora abbiamo un Governo in proroga; forse qualcuno voleva prorogare valutando *a posteriori* la precedente legislatura, che è finita tre mesi fa o, comunque, si è conclusa con l'atto elettorale di tre mesi fa

Le due modifiche apportate dalla Camera appaiono due toppe peggiori del buco. La prima modifica, come è stato fatto notare, pone un limite, il 30 settembre. Noi avevamo proposto un altro limite, ancora più breve; ma il problema è il limite del 30 settembre, già a detta degli stessi commissari, sarà ulteriormente superato a fronte del fatto che non è detto che vi sia un Governo capace di fare delle nomine entro il 30 settembre, che siano poi approvate dai due terzi delle rispettive Commissioni, con una maggioranza parlamentare che si prefigura diversa da quella che, verosimilmente, sarà espressa da un Governo - semmai ci sarà in queste settimane. Pertanto, la toppa è peggiore del buco: mettendo la toppa di un limite, nell'incertezza del quadro politico che si sarà nel frattempo determinato, di proroga su proroga, avete posto un limite che voi stessi sapete sarà superato; con un altro decreto?

Proprio per queste ragioni noi crediamo che questo non possa essere un voto tecnico, ma che debba essere un voto di denuncia politica rispetto alle condizioni straordinarie di un regime di proroga che emerge in tutta evidenza oggi, ma che si configura come una proroga politica, che noi non possiamo accettare. Per questo esprimeremo un

Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Morando, onorevole relatore Cioffi, vorrei ringraziare i colleghi del Gruppo Partito Democratico che sono intervenuti,

Oggi la velocità di innovazione e di trasformazione dei mercati è più elevata nell'energia che negli altri settori. Prova ne è anche l'attenzione prioritaria dedicata dall'Unione europea a questo settore, con le nuove iniziative legislative: penso al nuovo pacchetto Clean Clean Energy for All Europeans. assicurando allo stesso tempo una rafforzata tutela dei consumatori. Ciò favorisce, peraltro, scelte di investimento efficienti e commisurate alle esigenze dei clienti. In questo contesto il regolatore (in questo caso ARERA), presidio tecnico e indipendente dei settori regolati, deve garantire che il cambiamento sia indirizzato a beneficio dell'interesse pubblico, mentre le scelte di politica energetica sicuramente sono e devono restare una prerogativa della politica. Al regolatore la responsabilità di individuare gli strumenti e le modalità attuative più idonee. Nell'attuazione di questo delicato compito, la legittimità del regolatore deve trovare fondamento nella sua terzietà rispetto ai diversi soggetti portatori di interesse, nella chiarezza del mandato, in forme trasparenti di partecipazione diffusa alle decisioni. L'ARERA deve essere in grado di rispondere in modo efficace alle sfide, di consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli e informate, di permettere lo sviluppo di nuove forme *smart* di consumo, di trovare forme più efficaci per tutelare i i consumatori più vulnerabili, particolarmente esposti nel processo di liberalizzazione del mercato energetico. Vorrei sottolineare come la povertà energetica rappresenti già oggi un problema grave, destinato ad aggravarsi nel futuro a seguito delle difficoltà per molte famiglie di investire in efficienza energetica e rafforzare la verifica e il rispetto del quadro regolatorio. Un'ulteriore sfida per i prossimi anni è la gestione della quantità di investimenti necessari per la transizione verso un sistema energetico sostenibile (quella che viene chiamata economia circolare).

che ci porterà a nuove modalità di trasporto, dall'auto elettrica all'idrogeno; a nuovi modelli di consumo e di interazione tra consumatori; allo sviluppo di reti più intelligenti e flessibili. Su questo quadro regolatorio avrà quindi sempre più potere il livello sovranazionale e il livello europeo, dove opera un'agenzia europea istituita nel 2009, e quindi la nostra Autorità nazionale è a far sentire la sua voce nell'ambito di un contesto europeo importante, nell'ambito dell'Agenzia europea della regolazione, nell'ambito delle linee guida della Commissione europea. Questo è un pezzo della sfida più generale che abbiamo davanti. Stare in Europa, rafforzare l'integrazione europea e rafforzare politiche comuni anche sul tema dell'energia, ma sapendoci stare e salvaguardando l'interesse dell'Europa mediterranea.

misura che oggi si delinea come indifferibile e urgente per non privare il Paese di un organismo regolatore del sistema tariffario nazionale. L'Agenzia è nata nel 1995 con il nobile intento di evitare che i cittadini consumatori italiani continuino ad essere ulteriormente vessati e tassati su temi importantissimi come l'energia elettrica e il gas. Nel corso degli anni si sono aggiunti temi vitali come la gestione dell'acqua pubblica e i rifiuti; temi sicuramente molto delicati, visto che abbiamo a che fare con i servizi essenziali e soprattutto con le tasche dei cittadini.

Per quanto riguarda la gestione dell'energia elettrica, noi del Gruppo della Lega riteniamo debba essere a livello nazionale, anche perché in parte l'energia elettrica, purtroppo, siamo costretti a importarla dall'estero, quindi una gestione a livello nazionale ci sembra più che giustificata. Lo stesso dicasi per il gas: ne produciamo pochissimo e ne abbiamo pochissimo nel nostro sottosuolo per questo siamo costretti ad importarlo quasi totalmente dall'estero; quindi, anche su questo tema crediamo che una regia a livello nazionale sia assolutamente condivisibile. È invece estremamente importante e delicato il ragionamento sull'acqua, perché si tratta di un risorsa che ha chiaramente e indiscutibilmente una natura di bene

Infatti, nonostante il quesito referendario non abbia assolutamente inciso direttamente né sull'indizione delle gare, né sulla qualificazione di rilevanza economica del servizio idrico, il risultato referendario, avendo stabilito chiaramente l'assenza delle possibilità della remunerazione del capitale investito, fa venire meno - purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, ma noi alla fine riteniamo anche per fortuna - l'interesse degli imprenditori privati, che non hanno assolutamente la possibilità di fare degli utili sulla La gestione dell'acqua, per ovvie ragioni, è qualcosa che esisteva ben prima dell'entrata in funzione di ARERA, gran parte del territorio nazionale si gestiva tranquillamente questo servizio senza alcun problema particolare.

Ogni amministrazione pubblica locale ha sempre cercato, per ovvie ragioni, di gestire al meglio la propria acqua, assolutamente indispensabile per le famiglie e per i cittadini. Il Gruppo della Lega ritiene che l'eccessiva centralizzazione del servizio e della gestione, probabilmente con ulteriori oneri di struttura assolutamente non giustificati, sia esattamente quello che non deve essere fatto: non è l'economia di scala la priorità

si ipotizza anche lontanamente che vi sia un inquinamento all'interno delle reti di acqua pubblica. Chiaramente, la qualità dell'acqua passa attraverso forti investimenti sulle reti e sulle fonti idriche di approvvigionamento. La posizione della Lega è stata da sempre diretta a confermare che l'acqua è un bene pubblico, che le reti sono un patrimonio pubblico appartenente ai Comuni, che le gestioni efficienti e virtuose vanno garantite e tutelate, gli affidamenti *in house*, se possibile. Abbiamo sempre preferito la gestione pubblica dell'acqua, piuttosto che il monopolio dei privati o dei *partner* europei. Stessa cosa per i rifiuti, dove ARERA potrebbe essere utile per convincere molti territori - lo dico in maniera positiva - del Centro e del Sud Italia, dove spesso ci sono ancora amministrazioni locali reticenti in materia di raccolta differenziata e gestione corretta dei rifiuti. Dobbiamo ricordare e sottolineare che in Italia vi sono territori, in gran parte concentrati nella parte settentrionale del Paese, dove la questione è stata affrontata da tempo in maniera assolutamente adeguata, tanto che, non da adesso ma già da parecchi anni, gli obiettivi che anche a livello europeo sono stati fissati per il nostro Paese sono già stati raggiunti e abbondantemente superati.

Un Paese, il nostro, dove ci sono territori che in maniera virtuosa raggiungono livelli straordinari di efficienza. Lo dico solo a titolo di esempio. Ci sono territori che raggiungono anche l'85 per cento di raccolta differenziata. Abbiamo luoghi dove le tariffe per una famiglia famiglia media di quattro persone non superano i 200 euro all'anno. Altresì, vi sono territori dove le stesse persone, con le stesse dimensioni del nucleo familiare e della casa, pagano tariffe pari a più del doppio. Per quattro Non è possibile

Abbiamo in Veneto (cito esempi anche in Friuli e Lombardia) situazioni impiantistiche di eccellenza, che trasformano tutto il rifiuto in risorsa. Ci sono aziende che trasformano la frazione organica dei rifiuti completamente in energia, passando ad esempio attraverso il biometano, che viene usato per far funzionare gli automezzi. Pensiamo - non è fantascienza - che dal biometano si riesce a estrarre (in termini tecnici si dice strippare) la CO2 che viene usata anche nel settore alimentare. Ci sono aziende che trasformano i rifiuti in acqua calda con il teleriscaldamento, aziende che trasformano i rifiuti in elettricità per le case e per gli impianti stessi, aziende aziende che trasformano i rifiuti in *compost* o terriccio per l'agricoltura o il florovivaismo. Questi sono esempi che dobbiamo prendere in considerazione

Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo di Forza Italia annuncia il proprio voto favorevole. Ci troviamo di fronte a un provvedimento necessario, direi quasi dovuto. Anche noi confermiamo, da un punto di vista tecnico, una presa d'atto del fatto che i componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, cosiddetta ARERA, che durano in carica sette anni e non possono essere confermati, sono arrivati alla loro scadenza naturale, la terza consiliatura. E opportunamente, con delibera 8 febbraio 2018, il collegio di ARERA, in vista dell'approssimarsi della suddetta scadenza, ha stabilito di conformarsi al parere del Consiglio di Stato e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del proprio mandato, stabilendo altresì che in detto regime di *prorogatio* il collegio medesimo esercita le proprie funzioni solo limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. Va ricordato che il parere del Consiglio di Stato, al quale si era conformata anche la seconda consiliatura dell'Autorità, ha affermato in sintesi che l'Autorità, in quanto istituzione indipendente di nomina anche parlamentare e non soggetta, in caso di vacanza dell'organo, al potere sostitutivo del Governo, è sottratta dall'applicazione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. che prevede la *prorogatio* di quarantacinque giorni degli organi amministrativi. Considerata la particolare rilevanza e la non surrogabilità delle funzioni affidate all'Autorità, nel caso di simultanea scadenza di tutti i componenti del collegio della medesima Autorità, si deve ammettere, a titolo eccezionale, la possibilità di una specifica *prorogatio*, al fine di assicurare la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo collegio. Tale specifica *prorogatio* si deve tuttavia esaurire entro il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, di sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del mandato, con limitazione però dei poteri e degli atti di ordinaria amministrazione da quelli indifferibili e urgenti. Con delibera 9 aprile 2018 il collegio dell'Autorità, a fronte del contesto congiunturale determinatosi a seguito delle elezioni politiche, nel quale tutt'ora il quadro delle istituzioni competenti al procedimento di nomina dei componenti dell'Autorità stessa risulta ancora incompleto, e in mancanza di interventi legislativi indicanti la prosecuzione o la reintegrazione la prosecuzione o la reintegrazione dell'esercizio delle funzioni da parte della terza consiliatura, ha precisato che, concluso in data 12 aprile 2018 il periodo di specifica *prorogatio* della terza consiliatura dell'Autorità, a decorrere dal giorno 13 aprile 2018 e sino l'insediamento della prossima quarta consiliatura, in assenza di interventi di altre istituzioni che indichino nelle more la prosecuzione e il reintegro dell'esercizio delle funzioni da parte dell'attuale consiliatura, l'attività amministrativa dell'Autorità sarà curata dagli uffici della medesima, nei limiti delle funzioni Il giorno successivo è intervenuto - come è noto - il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, che ha disposto l'estensione del periodo di specifica *prorogatio* del collegio dell'Autorità. Il decreto-legge ha consentito al collegio dell'Autorità la prosecuzione nell'esercizio delle proprie funzioni, sia pure nei limiti già individuati dal sopracitato parere del Consiglio di Stato, degli atti di ordinaria amministrazione o indifferibili e urgenti. È chiaro, peraltro, che tali provvedimenti, ancorché nulli, rimarranno efficaci fino a quando la nullità degli stessi non verrà accertata dal giudice amministrativo, in caso di eventuale mancata conversione del decreto-legge È per questa ragione quindi che, evidenziando rilevanti problemi di precarietà dei provvedimenti adottati sulla base di decreto-legge non convertito, offre serie argomentazioni - noi crediamo anche assolutamente non optabili - a supporto della necessità di conversione di questo decreto-legge, onde assicurare la certezza del diritto e la stabilità del quadro regolatorio. La vera novità è che l'Autorità si dovrà occupare anche della regolamentazione e del controllo del settore dei rifiuti. Su questa scelta credo che si aprirà un dibattito importante - io spero - nelle Aule parlamentari e nelle Commissioni competenti, per alcune materie che già sono state accennate, sulle quali evidentemente omettiamo una discussione in fase di dichiarazione di voto. Ma è chiaro che, nell'attività di regolamentazione e controllo del settore dei rifiuti, è necessario - lo diciamo chiaramente - che si operi, da un lato, nella direzione dell'economia circolare e, dall'altro, con regole aperte al mercato e alla concorrenza, consapevoli che ciò apre un dibattito e che dobbiamo coniugare il mercato e la concorrenza con un'eccellenza che abbiamo - come è già stato citato da alcuni colleghi - all'interno delle *multiutilities* che oggi si occupano di questi servizi nel nostro Paese che in molti casi, pur essendo quotate in borsa, sono a maggioranza pubblica. È chiaro che è necessario coniugare la presenza di eccellenze da un punto di vista pubblico con l'apertura al mercato per quel che riguarda il privato: solo l'apertura al mercato darà la possibilità ai cittadini di risparmiare sui costi dei servizi, a partire dalla tassa sui rifiuti.

Anche per queste ragioni la nomina del collegio dell'Autorità ha grande rilevanza - non lo devo né sottolineare, né evidenziare - e necessita - secondo noi - di un ampio consenso. Forza Italia vigilerà e sarà attenta perché i futuri membri abbiano i requisiti di alta professionalità richiesti e il nostro voto sarà favorevole e soprattutto perché - e concludo - le aziende e i consumatori possano avere nell'Autorità un presidio autorevole.

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame è un atto dovuto, che reca misure urgenti al fine di assicurare la continuità delle funzioni di ARERA attraverso la proroga della durata in carica dei rispettivi componenti il collegio, nominati per sette anni, con decreto del Presidente della Repubblica 2011 e scaduti l'11 febbraio 2018. Faccio una prima considerazione: non saremmo qui oggi se fosse stato accolto l'emendamento che avevamo presentato alla legge

Il decreto- legge è composto da due articoli, nel primo dei quali si dispone che i componenti continuino a esercitare le proprie funzioni per gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità, non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018. Esso stabilisce che durante questa *prorogatio* l'ARERA trasmetta alle Camere una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti. Inoltre prevede che, nella prima relazione, vengano esposte le motivazioni degli atti adottati nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto-legge fino alla sua ratifica. L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento. È quasi inutile sottolineare l'importanza che riveste l'Autorità, a cui spetta il compito di definire il quadro regolatorio nell'ambito di settori primari come energia, acqua e rifiuti; ambito regolatorio che va però definito in base a dei principi stabiliti dal Parlamento. Ad essa spetta, in particolare, promuovere una sana concorrenza, l'efficienza e adeguati sistemi tariffari, con l'obiettivo di consolidare in tutto il Paese elevati *standard* di qualità dei servizi al miglior prezzo possibile per i cittadini.

però è un ruolo che non sempre è stato rispettato, anzi spesso non è stato rispettato. Molte volte - come ricorderanno i colleghi della scorsa legislatura, il Movimento 5 Stelle ha denunciato in quest'Aula e in altre sedi, con ogni mezzo,

oltrepassato le sue facoltà; provvedimenti che hanno ostacolato o addirittura si sono posti contro gli indirizzi dettati dalle norme approvate dal Parlamento.

per la fornitura di energia elettrica, con il relativo superamento della progressività, che ha comportato l'incremento di quasi 100 euro all'anno della bolletta per milioni di clienti domestici, quelli che consumano poca energia e spesso rappresentano le famiglie più deboli.

per la realizzazione di interventi sia di risparmio energetico e di efficienza energetica, che di autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile. Viceversa, questa riforma ha favorito la creazione di rendite dei distributori di energia. In questo caso, quindi, l'Autorità ha esercitato un potere che non gli compete e ha determinato l'indirizzo di politica energetica nazionale, politica energetica nazionale che invece spettava e spetta a noi, al Parlamento. Ora è chiaro che, rispetto a qualche mese fa, la composizione parlamentare è cambiata e quindi il Movimento 5 Stelle si augura che il Parlamento si riprenda le proprie prerogative. massimo rispetto per quelle dell'Autorità, ma il Parlamento deve riprendersi le proprie esclusive prerogative parlamentari, e il termine «esclusive» significa moltissimo.

si è svestito del proprio ruolo e lo ha lasciato in mano all'Autorità. Noi, invece, dobbiamo riprenderci questo ruolo perché afferisce a servizi essenziali come acqua, energia e rifiuti. Attenzione, perché dalle regole che l'Autorità determina non dipende solo il rispetto dell'indirizzo politico parlamentare e degli accordi internazionali su clima e energia ma, in soldoni, le opportunità sociali, ambientali ed economiche che l'attuazione di queste politiche crea verso la collettività. Ho detto pochi minuti fa che la riforma della tariffa ha

Questo significa che il ruolo dell'Autorità è importantissimo e può determinare quanto andremo verso nuovi modelli sostenibili decarbonizzati, quanto andremo verso una transizione energetica rinnovabile e verso l'economia circolare, quanto, quindi, avremo benefici interni diretti, capaci di stimolare la domanda interna, la crescita e il progresso economico in settori produttivi nazionali. Ricordo che abbiamo abbondanza di studi che quantificano in mezzo milione - come saldo complessivo, quindi tenendo conto anche delle perdite - i nuovi posti di lavoro che possiamo creare abbracciando efficienza energetica e fonti rinnovabili. Ma, attenzione, questo risultato non lo raggiungiamo se non c'è un'efficace e soprattutto rapida stesura delle regole Noi corriamo il serissimo rischio di perdere ulteriori posti di lavoro. Come ricordate tutti, nelle fonti rinnovabili abbiamo perso 120.000 posti di lavoro negli ultimi sette anni;

afferisce a un milione di posti di lavoro. Tutta la filiera estesa della mobilità conta un milione di posti di lavoro. al mercato delle auto elettriche di circolare a pieno titolo, di entrare nel settore della mobilità, di entrare, soprattutto, nel mercato dei servizi elettrici perché, forse qualcuno non lo sa, negli altri

come fattore generatore di reddito per gli operatori. Voglio dire che nel futuro gli operatori non faranno più i soldi producendo elettricità, ma con il mercato del dispacciamento. Ora, capisco che sia un argomento un po' tecnico, che, magari, qui non tutti lo conoscono e che non è semplicissimo, ma noi siamo qui per anticipare e regolamentare il futuro, non per farci travolgere dal futuro e subirlo! *(Applausi dal La situazione politica attuale, ovviamente, non favorisce questo percorso. Quindi, come Movimento 5 Stelle, noi siamo assolutamente vogliosi e desiderosi di far partire questo Governo, di far partire le Commissioni e di lavorare in maniera tale che, finalmente, si possa nominare il nuovo collegio, introducendo figure naturalmente di grande competenza e professionalità nel settore, ma introducendo, decisamente, una discontinuità rispetto al comportamento tenuto nel precedente settennato, che ha comportato quei 120.000 posti di lavoro persi e, in questo momento, il rischio di perderne di ulteriori. Ai sensi della legge del 14 novembre 1995, i componenti dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministeri competenti che, in questo caso, saranno i sviluppo economico e dell'ambiente. Queste designazioni, però, sono previamente sottoposte al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti votato, come sapete, con la maggioranza qualificata dei due terzi: questo può avvenire ed è nostra responsabilità farlo avvenire, ma solo nel caso di un Governo pienamente legittimato, quindi di un Parlamento pienamente funzionante e di un Governo pienamente legittimato. Che non si pensi, invece, di fare manovre strane con Governi non pienamente legittimati, questo assolutamente non lo vogliamo permettere.

finestra"). Essendo concluso l'esame degli argomenti previsti dal calendario dei lavori, la seduta di domani, giovedì 31 maggio, non avrà luogo. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Il Senato è convocato a domicilio. La seduta è tolta